L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

è morto poche ore fa Massimo Bordin, la voce di Radio Radicale, così familiare a tutti noi e e a tanti italiani ascoltatori che lo hanno seguito ogni mattina, con la sua imperdibile rassegna stampa, che l'hanno seguito sugli speciali giustizia, su corrispondenze di vario tipo, dagli Stati Uniti, da Israele; Massimo Bordin, la voce della radio che ha anche e a lungo autorevolmente diretto. La La sua scomparsa ci ricorda quanto Radio Radicale ha rappresentato per l'intera informazione politica italiana, e non solo per quella audiovisiva, dalla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso fino ad oggi.

A noi resta il rimpianto per la sua malattia e la sua morte, dunque un cordoglio sentito ai familiari e alla redazione tutta. Sono convinta che questo Senato troverà modo di ricordarlo in maniera più adeguata di quanto possa fare io in modo così sommario in questo momento. Se ne va Massimo Bordin, se n'è andato: che la terra gli sia lieve; ma se ne va anche una parte di tutti noi.

Signor Presidente, tenevo ad associarmi al ricordo di Massimo Bordin. Lo dico con il massimo rispetto umano e professionale per l'attuale direttore Alessio Falconio, ma per me Massimo era Radio Radicale ed era la politica. Cominciare tutte le giornate, da quando la politica per me è diventata un interesse, ascoltando la rassegna stampa condotta da Massimo Bordin, era il modo per cominciare con la politica. Non era solo una rassegna stampa, era un'occasione di analisi, idee e approfondimenti. Massimo era un vecchio del mestiere e, come pochi, aveva cultura politica. È il caso di dire che si tratta di uno di quei vuoti che difficilmente possono essere colmati. Ritengo simbolicamente emblematico il fatto che

nelle parole che con grande emozione ha pronunciato la senatrice Bonino. Credo che sia davvero opportuno programmare un'iniziativa che ci permetta di raccontare bene e in profondità quanto grande sia stato il contributo che Massimo Bordin ha dato al giornalismo civile in Italia. sottolineare, in questo pochissimo tempo che mi è concesso, che la rassegna stampa mattutina di Massimo Bordin è stata, per non pochi italiani, un esercizio di educazione intelligente ai doveri e ai diritti di cittadinanza: non è stata solo il racconto di ciò che era scritto sui giornali, ma un modo per avere ragioni per non seguire un approccio semplicistico e demagogico al dibattito politico. A ispirarla era il principio che per ben orientarsi politicamente e ben decidere è necessario conoscere; e si conosce bene soltanto se si fa un confronto non fazioso tra le tante opinioni che naturalmente sono in campo, in una democrazia pluralistica come la nostra. Da questo punto di vista, è stato davvero un giornalista eccellente e a me fa particolarmente piacere ricordare anche non solo il Massimo Bordin autore della rassegna stampa mattutina, ma il corsivista

false di un giustizialismo illiberale, culturalmente subalterno e demagogico, che a mio avviso ha fatto tanto male alla democrazia di questo Paese. Bordin questa battaglia l'ha fatta con sobrietà, convinzione, grande vigore ed energia e dando davvero un contributo significativo. Ritengo che per queste ragioni si debba prevedere un'iniziativa che lo ricordi adeguatamente, anche a distanza di tempo da un evento che ci turba tutti in

mi unisco alle parole di cordoglio e affetto verso la famiglia le persone che erano vicine a Massimo Bordin. La sua rassegna stampa mi ha fatto compagnia la mattina per tanti anni, anche quando espletavo altre funzioni, quelle di magistrato, perché non era una mera lettura dei giornali, ma un modo di trattare le notizie della politica e della cronaca con ironia, con commenti che davano risalto alle notizie e con una passione politica che ho avuto modo di apprezzare anche personalmente, da Presidente del Senato, in occasione di incontri

cari quel tentativo di ricerca delle pagine dei giornali, quel dare valore alla notizia in relazione alla pagina in cui era stata collocata dalle redazioni e una serie di particolari della sua attività che lo rendevano unico ai miei occhi. A nome del Gruppo di Liberi e Uguali, mi unisco quindi al cordoglio nei confronti dei familiari

nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea,

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, la Commissione finanze ha concluso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 2019, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito in caso di un recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Il lavoro in Commissione è stato positivo, equilibrato e spesso condiviso. Ringrazio i senatori, per il loro contributo e per l'andamento scorrevole e celere dei lavori, lavori, nonché i funzionari della Commissione per il loro fondamentale ruolo tecnico. Il decreto-legge è stato emanato in un momento in cui vi è ancora incertezza sui tempi e sulle modalità di uscita dall'Unione europea del Regno Unito, che ha raggiunto un accordo di recesso il 22 novembre 2018, il quale tuttavia è stato respinto dal Parlamento del Regno lo scorso 29 marzo 2019, data coincidente con la scadenza del biennio dalla notifica della determinazione di recedere. Nel Consiglio europeo straordinario svoltosi il 10 aprile 2019, dedicato a valutare le modalità con le quali il Regno Unito intende procedere in seguito alla mancata approvazione dell'accordo di recesso, ha adottato conclusioni nelle quali, in particolare, sulla sulla base delle richieste del Regno Unito ha concordato di concedere un'ulteriore proroga del termine *ex* articolo 50 del Trattato dell'Unione europea per consentire la ratifica dell'accordo di recesso. Tale proroga, in ogni caso, non potrà andare oltre il 31 ottobre 2019, né dovrà consentire di minare il regolare funzionamento delle istituzioni dell'Unione europea. È stato stabilito, inoltre, che durante il periodo di proroga il Regno Unito rimanga stato membro dell'Unione europea con pieni diritti ed obbligazioni e possa revocare la notifica del recesso in qualsiasi momento. Le disposizioni in esame affrontano principalmente l'esigenza di fornire un quadro giuridico chiaro ai rapporti finanziari tra Italia e Regno Unito. A queste se ne aggiungono alcune che, pur non essendo direttamente connesse alla Brexit, sono volte a garantire la sicurezza dei cittadini e la stabilità finanziaria. Il capo I, all'articolo 1, novella il decreto-legge n. 21 del 2012, recante «norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni». In particolare, la norma è volta ad aggiornare la disciplina in materia di poteri speciali, in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. Tali poteri sono assistiti da un obbligo di notifica applicabile alle parti contraenti di contratti o accordi che consenta all'Esecutivo il tempestivo esercizio del veto. Nel capo II il decreto-legge realizza uno scenario in cui ai soggetti italiani che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo, viene consentito, salvo diversa previsione del Regno Unito, di proseguire l'operatività, mentre agli operatori del Regno Unito viene imposto un restringimento del campo d'azione parziale (banche, imprese d'investimento e istituti di moneta elettronica) o totale (istituti di pagamento, fondi e relativi gestori e imprese di assicurazione). In particolare, infatti, l'articolo 2 reca la disciplina transitoria applicabile per garantire la stabilità finanziaria in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e fornisce le definizioni di alcune espressioni utilizzate nel testo del decreto-legge, come quella delle imprese bancarie, finanziarie e assicurative destinatarie delle norme. L'articolo 3 disciplina la continuazione, durante il periodo transitorio, dell'attività da parte di banche, imprese d'investimento e istituti di moneta elettronica già autorizzati alla prestazione dei relativi servizi. La possibilità di continuare ad operare è condizionata alla notifica alle autorità competenti e alla presentazione di un'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività entro sei mesi dalla data di recesso. La disciplina distingue i soggetti che operano su base stabile, avvalendosi del diritto di stabilimento, da quelli che operano in regime di libera prestazione. In questo secondo caso, ferma restando la necessità di notifica, sono escluse le seguenti attività: per le banche, la possibilità di effettuare la raccolta del risparmio; per le imprese d'investimento, la possibilità di operare nei confronti dei clienti al dettaglio. Per l'istituto di moneta elettronica, invece, è esclusa *in toto* l'operatività in regime di libera prestazione dei servizi. L'articolo prevede, poi, due regimi speciali di prosecuzione dell'attività: per le banche e le imprese d'investimento del Regno Unito abilitate alla partecipazione all'asta dei titoli di Stato alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che possono continuare a svolgere i servizi e le attività bancarie, ad eccezione dell'attività di raccolta del risparmio, nonché i servizi e le attività d'investimento senza necessità di notifica; uno per la gestione degli eventi del ciclo di vita di particolari categorie di contratti derivati *over the counter* in essere alla data del recesso. Durante l'esame, è stato approvato l'emendamento 3.2, volto a chiarire che le banche e le imprese d'investimento operano secondo quanto previsto dal TUB e dal TUF fino al giorno antecedente al recesso. L'articolo 4 elenca invece i soggetti del Regno Unito operanti in Italia che sono tenuti a cessare l'attività entro la data di recesso: istituti di pagamento, gestori di fondi, organismi d'investimento collettivo del risparmio, istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati. Devono altresì cessare la raccolta del risparmio e la prestazione dei servizi di investimento, qualora effettuati in regime di libera prestazione dei servizi, senza una stabile organizzazione sul territorio della Repubblica. Nell'elenco rientrano inoltre i soggetti autorizzati a proseguire l'attività che non abbiamo notificato l'intenzione di farlo all'autorità e che non prestino un'istanza di autorizzazione trascorsi sei mesi dall'inizio del periodo transitorio. Al fine di garantire maggiore trasparenza e tutelare la clientela, è stato previsto un obbligo di comunicazione in capo ai soggetti che cessano le suddette attività, volto a garantire la cessazione delle stesse. L'articolo 5 indica i soggetti italiani per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio. La prosecuzione viene condizionata ad obblighi di notifica alle autorità competenti e alla presentazione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento delle relative attività entro i dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio. Tali adempimenti, comunque, non sono necessari se i soggetti hanno presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti entro la data del recesso, come previsto dall'emendamento 5.1. L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiana (ad esempio, Borsa Italiana SpA) possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e che, viceversa, i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica. Tale facoltà viene riconosciuta subordinatamente alla presentazione, entro la data del recesso, di un'istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito da parte dei gestori italiani e, viceversa, di una in Italia da parte dei gestori del Regno Unito. L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese d'investimento e gli istituti di pagamento e di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con le clientele disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dall'articolo 128-*bis* del TUB e, per quanto riguarda quelli d'investimento, dall'articolo 32-*ter* del TUF. L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere le attività e i servizi bancari e d'investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e d'indennizzo degli investitori. di diritto si applica anche ai soggetti che operano nel regime di libera prestazione di servizi, ai gestori di fondi, alle banche e alle imprese d'investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto all'articolo 4, salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema italiano (di garanzia o indennizzo) una dichiarazione di quello del Regno Unito, attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. Vengono, inoltre, stabiliti obblighi informativi nei confronti dei depositanti e degli investitori, che consentono loro di essere correttamente informati sulle tutele loro applicabili. L'articolo 9 è relativo al settore assicurativo e dispone la cancellazione delle imprese di assicurazione del Regno Unito operanti nel territorio della Repubblica, in regime sia di stabilimento sia di libera prestazione dei servizi, dall'elenco delle imprese dell'Unione europea dopo la data di recesso. Nel periodo transitorio le imprese di assicurazione del Regno Unito proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti in essere e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Ai sensi del successivo articolo 10, anche gli intermediari assicurativi o riassicurativi del Regno Unito, ossia i soggetti attivi nella distribuzione di polizze assicurative operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso e sono cancellati dal relativo registro. Per tutelare i clienti, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. L'articolo 11 dispone invece la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. L'articolo 12 prevede che i fondi d'investimento del Regno Unito siano assimilati a quelli europei per tutto il corso del periodo transitorio. Si consente pertanto ai fondi pensione italiani di continuare ad investire in fondi del Regno Unito. L'articolo 13 reca una disposizione di carattere generale e dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso raggiunto il 22 novembre 2018. In particolare, è previsto che fino al 31 dicembre 2020 si continuino ad applicare ai soggetti del Regno Unito che operano in Italia le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea. Gli articoli 14, 15, 16 e 17 contengono norme nelle seguenti materie: soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; concessione della cittadinanza italiana ai cittadini del Regno Unito; potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito; prestazioni sanitarie e di sicurezza sociale nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale. In materia aeroportuale è stato approvato l'emendamento 17.0.1, volto a conservare l'esistente sistema tariffario aereo tra l'Italia e il Regno Unito, in attesa dell'eventuale Brexit, al fine di scongiurare l'aumento delle tariffe che deriverebbe dalla perdita dello *status* comunitario al secondo Paese. È stata inoltre introdotta una disposizione che, a condizione di reciprocità, salvaguarda salvaguarda la posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito presenti in Italia alla data del recesso o che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020. L'articolo 18 autorizza la sottoscrizione di quote di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) da parte dell'Italia, per un ammontare pari a circa 6,9 miliardi di euro. La sottoscrizione dell'Italia è resa necessaria per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale del Governo. È prevista la facoltà di assunzione di personale da parte del connessa alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei e internazionali in materia economico-finanziaria. Durante i lavori sono state introdotte due disposizioni riguardati i principi contabili internazionali, in particolare l'emendamento 19.0.3 e l'emendamento 19.0.4. Un'altra importante novità riguarda la possibilità, per la Cassa depositi e prestiti e le equivalenti strutture europee, di svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. titoli di Stato. In conclusione, al capo III, gli articoli da 20 a 23 del decreto-legge consentono la prosecuzione delle misure di supporto allo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, tramite la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza. A tal fine, si utilizzano i meccanismi disciplinati dal decreto-legge n. 18 del 2016, cui sono apportate alcune modifiche. Viene confermata la disciplina secondo la quale possono usufruire della garanzia dello Stato solo le cartolarizzazioni cosiddette *senior*, ossia quelle considerate meno rischiose, e non si può invece procedere al rimborso dei titoli più rischiosi, se prima non sono integralmente rimborsate le *tranche* di titoli coperti dalla garanzia di Stato. Le garanzie possono essere chieste dalle banche a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Si prevede che il prezzo della garanzia sia di mercato, al fine di non dar vita ad aiuti di Stato, e crescente nel tempo, allo scopo di tener conto dei più elevati rischi connessi a una maggiore durata dei titoli e d'introdurre nel meccanismo un incentivo a recuperare velocemente i crediti. Al fine del rilascio della garanzia, i titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono avere preventivamente ottenuto un *rating* uguale o superiore al *rating* BBB da un'agenzia di *rating* indipendente e inclusa nella lista di quelle accettate dalla BCE, secondo i criteri che le stesse sono tenute ad osservare.

Internet e vede la centralità dell'intelligenza artificiale, non solo per migliorare la produttività del nostro Paese, ma proprio per riposizionarne il modello industriale

nel periodo tra il 2016 e il 2025. Stiamo discutendo tanto di come far crescere il PIL nel Paese e i dati non sono confortanti: perché non fare un ragionamento approfondito

che i tre macrofenomeni della globalizzazione, dell'immigrazione e della digitalizzazione, che hanno una portata internazionale, non siano stati ben governati a livello europeo e non possano essere governati da un singolo Paese. Tornando alle tecnologie digitali,

Cari colleghi, non si può fare niente in tal senso: il digitale e il reale sono talmente permeati tra loro

poi si è unita la finanza come fattore di sviluppo di un Paese. Oggi dobbiamo iniziare a parlare anche di dato centrale nell'economia reale, dato generatore di nuova ricchezza, intorno al quale andiamo a costruire un pezzo importante del nostro PIL.

Negli ultimi due o tre anni abbiamo generato l'80-90 per cento dei dati rispetto al totale di quelli generati dall'inizio dell'umanità fino a un biennio, triennio fa (vale a dire, solo il 10-20

asse. Mettiamoci dentro, incuneiamoci lì. Noi abbiamo un *player* che è stato molto importante, il cui *brand* è ancora oggi mondiale; lo dico veramente, non solo per appartenenza al territorio, ma perché ci credo davvero. *(Richiami del Presidente).* Termino. Questo *brand* è Olivetti. Gli stabilimenti industriali Olivetti possono diventare veramente la sede di una piattaforma digitale europea,

tecnologia 5G. Credo tuttavia che sia il caso di aggiungere, perché è una questione rilevante, visto che si vuole parlare anche di sicurezza,

forse andrebbero lette con maggiore attenzione le indicazioni che vengono date nei documenti di sicurezza nazionale, che ogni parlamentare ha avuto

in modo sintetico ma puntuale, dal relatore, su come sistemare i crediti deteriorati delle banche, tanto per intendersi, si traduca nella sostanza in un rischio che è trasferito non tanto allo Stato e ai fondi a garanzia, quanto a coloro che andranno a sottoscrivere

assolutamente incomprensibile, tenendo conto del tipo di politiche che le forze della maggioranza vogliono portare avanti. Il problema è che, di fatto, pur

Ciò significa che una banca può fare un'operazione in base alla quale cartolarizza i famosi debiti in sofferenza (che pesano nei bilanci delle banche): si emettono titoli che avrebbero come garanzia dei mutui, ma il rischio viene trasferito ai sottoscrittori finali delle obbligazioni,

dei mutui. Francamente, credo che una politica in base alla quale, da una parte, si va a raccontare che difendono i risparmiatori e, dall'altra, si mette in piedi un sistema in cui invece il risparmiatore rischia di trovarsi il prodotto prefabbricato dalla propria banca, con la certificazione delle

non sia in linea con quanto detto e proclamato in tutte le salse da questo Governo del cambiamento.

strumenti che possono consentire il perpetuarsi di questa impostazione. Tenete conto che la società civile, quella che chiamereste semplicemente il popolo, avveduto e che un po' conosce i meccanismi, si rende perfettamente conto che questa roba entra in circolo con tutta una serie di conseguenze che possono essere negative per i singoli. In conclusione, credo che ci voglia un po' più di chiarezza di idee, con riferimento alla questione del 5G, e un poco più di coerenza con riferimento alla tutela dei risparmiatori.

Signor Presidente, il decreto-legge sulla Brexit, che disciplina servizi bancari, finanziari ed assicurativi in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo, vede il Partito Democratico sostanzialmente d'accordo con le misure di salvaguardia in relazione ad alcuni settori problematici conseguenti al possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un *deal* predefinito. Il decreto-legge interviene, tra le altre cose, con una serie di garanzie per le attività degli operatori del Regno Unito attivi in Italia e per quelli italiani attivi nel Regno Unito. Riteniamo che si tratti di una norma ordinamentale, che consente all'ordinamento giuridico italiano di funzionare, permettendo di continuare a lavorare, a studiare, a investire, a farsi curare, in sostanza ad operare, sia agli italiani presenti nel Regno Unito, sia ai sudditi di Sua Maestà britannica che si trovano nel nostro Paese: tutto ciò in conseguenza della rottura della concordia comunitaria scaturita dall'uscita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal sistema dell'Unione europea. Le norme puntano sostanzialmente a permettere a banche britanniche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica, che operano mediante succursali del Regno Unito, di continuare la propria attività in Italia anche durante il periodo transitorio, che il decreto-legge prevede in diciotto mesi, previa notifica alle autorità competenti tre giorni prima della data della Brexit. Le banche britanniche, che svolgono attività di raccolta del risparmio, non possono concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti. Per le banche che partecipano alle aste dei titoli di Stato non è invece richiesta la notifica, ad eccezione dell'attività di raccolta del risparmio. Per poter continuare ad operare in Italia, anche dopo il periodo transitorio, o costituire un intermediario italiano, questi soggetti dovranno presentare un'apposita domanda entro sei mesi dall'avvio della transizione. Nel decreto-legge si rafforza inoltre il *golden power* sulla tecnologia 5G, anche dopo le polemiche seguite agli accordi con la Cina sulla nuova Via della Seta. La rete 5G è una struttura portante delle nostre infrastrutture digitali ed era quindi fondamentale e importante intervenire in questo ambito. Soprattutto a seguito degli accordi che si sono sviluppati con la Cina, il Governo ha deciso di inserire queste norme accanto a quelle preponderanti sulla Brexit. Con questa scelta l'operatore o gli operatori di telecomunicazione che vorranno acquisire le reti 5G dovranno comunicarlo preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri con un certo anticipo, affinché poi il Governo possa decidere se esercitare il veto sull'operazione oppure imporre specifiche prescrizioni. prescrizioni. Credo che sia quanto mai importante - ed era anche fondamentale farlo in maniera celere dopo l'accordo con la Cina - andare a normare questi delicati aspetti. in discussione regola anche le prestazioni sanitarie in caso di *no deal* per i cittadini britannici. Il testo prevede che, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, per quei soggetti si deve applicare fino a tutto il 2020 il regolamento europeo n. 883 del 2004 per le prestazioni sanitarie e sociali. Il decreto-legge prevede che le banche del Regno Unito, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica britannici operino in conformità alle disposizioni in materia bancaria e finanziaria, e siano loro applicabili loro applicabili dal giorno antecedente la Brexit. Questa previsione vale fermo restando quanto previsto dal decreto per il periodo transitorio. Una volta rilasciata l'autorizzazione, gli operatori potranno operare in via definitiva secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali applicabili, fermo restando quanto previsto per le istanze autorizzative per le banche e le imprese di investimento aventi sede nel Regno Unito e abilitate alla partecipazione alle aste di titoli di Stato, per i quali non è richiesta la presentazione della notifica, salvo che per continuare ad esercitare l'attività di raccolta del risparmio. Le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che alla data del recesso prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere in Italia le stesse attività solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali. Il decreto-legge stabilisce anche che deve svolgersi entro quindici giorni dalla Brexit l'obbligo di comunicare ai clienti, nonché agli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi alle autorità competenti, le iniziative adottate per garantire l'ordinata cessazione dell'attività da parte di quei soggetti del Regno Unito che operano nel territorio italiano e che per il decreto-legge dovranno appunto interrompere le proprie azioni in Italia entro la data della Brexit. Si tratta degli istituti di pagamento del Regno Unito, dei gestori dei fondi del Regno Unito, degli OICR, nonché degli istituti di moneta elettronica che operano sul territorio italiano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati, così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento in regime di libera prestazione a favore dei clienti al dettaglio. Sono ammesse dopo la Brexit le operazioni per la chiusura dei rapporti già in essere, ma nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso, con l'osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Entro sei mesi tali soggetti proseguono l'attività svolta precedentemente alla data della Brexit solo per la gestione dei rapporti in essere alla data di recesso, senza possibilità di concludere nuovi contratti né di rinnovare, anche tacitamente, quelli esistenti. Un'altra norma del decreto-legge prevede che i soggetti italiani che operano nel Regno Unito possano continuare le proprie attività dopo la Brexit nel periodo transitorio di diciotto mesi previa notifica alle autorità competenti nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito. Tale notifica va effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti alla Brexit. I soggetti italiani possono continuare ad operare nel territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio oltre il periodo transitorio se entro dodici mesi anteriori alla fine dello stesso periodo transitorio presentino alle autorità competenti un'istanza apposita. I soggetti italiani che abbiano già operato l'istanza entro la data della Brexit non saranno tenuti alla notifica prevista per operare nel periodo transitorio. Credo che l'azione che abbiamo svolto in Commissione di analisi degli emendamenti, anche con nostre proposte così come con il dibattito che abbiamo sviluppato su quelli presentati da altri colleghi, abbia permesso sicuramente di migliorare il provvedimento. Siamo soddisfatti del fatto che le norme relative al Comitato interministeriale per l'economia digitale siano uscite da questo provvedimento. Abbiamo detto che anche per noi questo aspetto è importante, è da trattare e da sviluppare, anche in coerenza con quelle che oggi sono le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica per il credito ed il risparmio e crediamo che ci debba essere un'altra sede nella quale poter discutere di queste specifiche ed importanti norme. Riteniamo importante e rilevante che si sia proceduto a eliminare le norme che avevano un'attinenza con l'operatività bancaria e, in modo particolare, con alcune tipologie specifiche di banche: erano norme intruse che siamo lieti siano state accantonate da questo provvedimento. Resta, invece, aperta - mi auguro che anche nella discussione generale che stiamo sviluppando possano esserci elementi positivi di novità - la questione relativa all'aeroporto

esserci e debba consentire a chi oggi gestisce il sistema aeroportuale lombardo di poter continuare a farlo nelle condizioni migliori possibili, tenuto conto di quanto sta

È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.

Leggendo la scheda di lettura, che il Senato invia a tutti i senatori relativamente agli atti che sono all'attenzione delle Commissioni e dell'Aula,

di lettura, all'articolo 1 ci sono l'oggetto e l'ambito di applicazione, ma in questa scheda di lettura l'oggetto e l'ambito di applicazione sono stati inseriti all'articolo 2.

con una fionda, all'ultimo minuto, nel documento della Brexit, che non c'entra assolutamente nulla con il provvedimento che oggi quest'Assemblea si accinge a votare. Non abbiamo posto questioni, se non quelle ricordate poco fa dai colleghi, sul provvedimento della Brexit. C'è qualche necessità di aggiustamento, ma l'elemento 5G, estremamente ben descritto poco fa dalla collega Tiraboschi,

sul 5G. L'Europa chiude questo canale - che riguarda anche l'Italia e che per noi vale circa 2,5 miliardi di euro

Noi abbiamo tentato di porre rimedio a questo e non lo dico perché è un problema di Forza Italia (se fosse un problema di Forza Italia si risolverebbe tutto), ma perché è un problema di questo Parlamento.

ci è stato chiesto un testo 2, dalla Commissione, e noi diligentemente abbiamo predisposto un nuovo testo, l'emendamento 1.11 (testo 2), abbiamo scritto che il gruppo di coordinamento di cui al comma 4 trasmetta trimestralmente una relazione nientemeno che al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Che vuol dire: il comitato vuole avere le mani libere? Lo dico a voi senatori: il comitato - e non quello parlamentare, ma il comitato che siede a Palazzo Chigi, che non è composto da rappresentanti della politica

si permette di entrare nel merito di queste questioni? Guai a voi parlamentari se vi interessate delle sorti del Paese, perché il comitato vuole avere le mani libere! Onestà

scatole nere, viene inserito con una fucilata all'interno di un provvedimento che non c'entra assolutamente nulla e parla di Brexit, che è un argomento altrettanto importante; viene esautorata la Commissione di merito; non ci viene consentito di discutere nel merito di questo argomento, soltanto la senatrice Tiraboschi ha sollevato con dovizia di particolari un argomento del genere e lei, a una nostra richiesta di inserire un controllo del Parlamento, dice: «Vogliamo le mani libere». Vi dovete vergognare!

gentili colleghi, questo decreto-legge pone soluzione ad un errore, un errore di presunzione o forse una sottovalutazione delle implicazioni che il voto sulla Brexit ha determinato. Ad oggi, abbiamo poche certezze e tanti dubbi: questo testo di legge di cui discutiamo è stato elaborato per fornire uno strumento utile ai tanti lavoratori, italiani e britannici, e alle tante aziende per contrastare la situazione di incertezza che verrebbe generata da una uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza la ratifica di accordi che ne limitino l'impatto. Parlo di sottovalutazione, potrei anche parlare di leggerezza per riferirmi al voto che i cittadini britannici hanno espresso nel giugno 2016, fomentati da forze politiche miopi che anche subodorando le difficoltà legate all'esito della vittoria di misura

Cosa resta, però, è il danno fatto alla Gran Bretagna e all'Europa tutta. Tra l'altro, un'uscita senza accordo è uno schiaffo molto forte a quasi la metà degli inglesi, cento dei cittadini, come dicevo poc'anzi, che si erano espressi in favore dell'Unione europea e che ora si vedono dimenticati totalmente dai loro rappresentanti politici. Rappresentanti che, ricordo, sono stati capaci in pochi giorni di votare contro un'uscita dall'Europa senza accordo, per tre volte contro l'accordo stesso, chiuso dalla *premier* May, e anche contro un nuovo *referendum* sulla Brexit. Praticamente è la resa delle armi di chi è stato chiamato a rappresentare gli elettori e deve prendere alcune decisioni, nel bene o nel male. Chi ne fa le spese? Ovviamente, tutti i cittadini, europei e britannici. I legami che abbiamo con il Regno Unito sono stretti e molto importanti per centinaia di aziende e professionisti. Il ruolo che Londra ha svolto in questi anni, come centro economico e finanziario di tutta Europa, ci pone ora di fronte alla necessità di ridefinire e riorganizzare l'intero mercato finanziario intra e extra europeo. In apertura del mio intervento parlavo di pochissime certezze che abbiamo in questa fase di transizione e purtroppo sono tutte certezze molto negative. Innanzitutto, parliamo del settore bancario e finanziario: già in questi ultimi due anni tutti i grandi gruppi bancari hanno dovuto ricollocare le loro sedi, spostare personale, spendere centinaia di milioni di euro per contrastare questa situazione. In secondo luogo, le persone: sono centinaia di migliaia gli europei che per lavoro si trovano nel Regno Unito e che vivono un periodo di estrema incertezza. Infine, gli scambi commerciali: come Paese abbiamo un *export* verso il Regno unito di oltre 23 miliardi di euro mentre importiamo merci per soli 11 miliardi. Un saldo commerciale di oltre 12 miliardi a nostro favore che purtroppo soffrirà di una contrazione per le nostre aziende, che patiranno sicuramente per questa situazione. Prevenire è meglio che curare. Quante volte lo abbiamo sentito dire? Proprio per questo è stato proposto il testo che stiamo discutendo oggi: per prevenire le implicazioni di una *hard* Brexit, perché dopo sarebbe troppo tardi. Se è pur vero che gli accordi principali sono coordinati a livello europeo, dotarci di strumenti flessibili per un periodo di transizione è quanto mai necessario. In particolare, verranno tutelati i gruppi bancari, gli intermediari e gli operatori, al fine di assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati e la tutela degli investitori e della clientela. Per i cittadini britannici residenti da almeno cinque anni nel nostro Paese si prevede la possibilità di richiedere uno speciale permesso di soggiorno, che consentirà la loro permanenza sul territorio italiano, contestualmente alla salvaguardia dei diritti sanitari e sociali. Giustamente vengono, dopo tanti anni di difficoltà organizzative, potenziati gli uffici consolari del Regno Unito, vista la mole di lavoro che li impegna ogni giorno. Onestamente, fatemi dire, è scandaloso che questo potenziamento forte degli uffici e del personale necessario a gestire le pratiche non sia stato fatto prima, dagli scorsi Governi. Gli italiani registrati in Gran Bretagna risultano essere oltre 330.000. Ma se contiamo quanti non sono registrati all'AIRE, il numero dei nostri connazionali arriva alle 700.000 unità. Un numero impressionante di persone a cui, fino ad oggi, non è corrisposto un egual impegno delle nostre istituzioni. Ma tornando al testo del provvedimento, voglio lanciare un campanello d'allarme. Qui mancano due elementi fondamentali, ma sono sicuro che il Governo li integrerà in provvedimenti futuri: il primo, è un incentivo per il rientro di tanti cittadini italiani che sono emigrati nel Regno Unito e che costituiscono un patrimonio di esperienza e di capacità che il nostro Paese deve valorizzare. Oggi ragioniamo su cervelli e ricercatori, ma dobbiamo allargare i nostri orizzonti. Per coloro che hanno maturato importanti esperienze lavorative all'estero, anche in assenza di un titolo di laurea, è nostro interesse che tornino nel nostro Paese ad arricchire il nostro tessuto lavorativo e produttivo. Il secondo elemento, non meno importante, è uno scudo per le tante aziende che esportano merci in Gran Bretagna. Il settore agroalimentare *in primis*, ma non solo. È necessario pensare preventivamente a norme fiscali per le tante realtà che certamente avranno sofferenze dalla Brexit, anche in presenza di accordi con l'UE. Concludo con una speranza. La mia opinione personale è che gli inglesi, se andranno al voto nelle prossime elezioni europee il 26 maggio, lo faranno per dare un segnale molto forte al loro Governo, un segnale di unità, un segnale europeista. Andranno in massa ai seggi per attribuire simbolicamente al 26 maggio la data del secondo *referendum*, quel *referendum* non ancora concesso e più volte richiesto dalla piazza. Ci sono molti modi per perdere la giusta via, ma solo uno per ritrovarla: tornare sui propri passi. Un anonimo scrisse: «Ci vuole coraggio per innamorarsi, ma ci vuole ancora più coraggio per tornare indietro e riparare quello che si è rotto». Ecco, io vorrei parafrasare questo anonimo: ci vuole coraggio per andarsene ma ci vuole ancora più coraggio per tornare indietro e ricostruire insieme una nuova Europa, che veda in questa grande comunità anche i cittadini inglesi. Possono ancora tornare sui propri passi e io mi auguro possano trovare quel coraggio che non aspetta altro di essere palesato.

un tema sul quale abbiamo perso tutte le certezze che avevamo. Pensavamo che gli inglesi fossero un popolo estremamente pratico, interessato a portare avanti l'interesse pubblico, con una programmazione chiara. Questi capisaldi del pensiero di noi italiani nel Regno Unito sono stati messi a dura prova dalla gestione della cosiddetta Brexit, della quale la storia ci dirà se è stato uno dei più grandi fallimenti del Dopoguerra da parte del Regno Unito o l'occasione per fare quel salto avanti che i proponitori della Brexit hanno venduto. Faccio notare che è ancora aperta la possibilità per il Regno Unito di guadagnare un'indipendenza nella politica commerciale, che potrebbe consentirgli, per esempio, di entrare in una zona di libero scambio, come quella nordamericana, estremamente efficiente, e di fungere da piattaforma per l'Europa in quel mercato. La presidenza Trump ha sempre sostenuto questa possibilità, che rimane uno degli argomenti forti della Brexit. Vedremo come andrà a finire. nella situazione in cui il Governo May si trova adesso, con la necessità di raccogliere consensi all'interno del Parlamento di Westminster, *across the aisle*, dall'altra parte, quindi nell'opposizione laburista, il principio della c*ustoms union*, dell'unione doganale, vale a negare questa possibilità. Quindi, ad oggi, nessuno ha certezze. Non si sa ancora se sarà quel grandissimo fallimento che viene venduto nei *media* internazionali o la possibilità di fare un salto in avanti. Ricordo che il Regno Unito è entrato nell'Unione europea, nel Mercato unico europeo, nel 1974, perché ha ritenuto che fosse commercialmente utile alle proprie imprese fare da caposaldo per imprese extraeuropee, in particolare quelle giapponesi, per farle entrare nel mercato europeo, che, nel frattempo, era diventato un esempio di successo. Non per niente, tutte le fabbriche giapponesi che sono arrivate in Europa si sono insediate nel Regno Unito. Dietro al pensiero dei *brexiteer,* cioè della fazione più dura (il cosiddetto *European* *reform* *group* del partito conservatore, c'è soprattutto questo obiettivo che, bisogna essere oggettivi, potrebbe essere anche una grande opportunità commerciale. Vedremo, la storia ci dirà da che parte sono andati. Quello che però è già nel presente e che dobbiamo valutare è che la Brexit, sinceramente, produce nel presente una serie di disastri.

Sulla base del principio di sovranità assoluta di quello che loro considerano un prestigioso e antico Parlamento nel mondo, quello di Westminster, i *brexiteer* hanno combattuto questa battaglia. Tuttavia, tutti noi abbiamo verificato che lo stesso Parlamento inglese, rispetto alla tradizione occidentale della divisione tripartita dei poteri da Montesquieu ad oggi, subisce una condizione

che solo adesso, dopo ben tre tentativi andati a vuoto del Governo di ottenere un'approvazione sull'accordo di uscita, viene scalfita; per cui adesso verifichiamo che il Governo inglese ha iniziato a rispettare un po' di più il Parlamento.

è determinato pertanto un problema di integrità del Regno Unito, con particolare gravità della situazione dell'Irlanda del Nord. Questo è stato esemplificato più volte attraverso il cosiddetto *hard border*, cioè il confine che si verrebbe a creare tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord e che gli accordi di pace oramai trentennali avevano cancellato. Quindi vedremo. Non siamo ancora in grado di decidere cosa succederà; verifichiamo che tutta una serie di principi che noi davamo per assodati sono saltati. Tra questi c'è, ahimé, la libertà di movimento all'interno dell'Unione europea. Quattro sono le libertà che gli inglesi hanno cercato di scalfire a Bruxelles e che invece i 27 Paesi hanno difeso, dimostrando che l'Europa, quando è unita, può essere estremamente efficace. Gli inglesi avevano sottovalutato la capacità di reazione e l'unitarietà della reazione degli europei e continuano, in certo modo, ancora a sottovalutata.

partite IVA e dei codici fiscali aperti a cittadini italiani da parte dell'autorità inglese: sono *national insurance number* attribuiti a cittadini italiani. Quindi vi sono effettivamente 700.000 cittadini italiani che si sono spostati nell'Unione europea liberamente, come hanno fatto in altri Paesi dell'Unione - vivaddio - ed è questo il grande successo dell'Unione europea, del disegno europeo. Troppe volte sottovalutiamo gli effetti positivi di far parte dell'Unione europea, compresa la libertà di movimento delle persone. è destinato a venire meno. Noi siamo stati molto generosi, con questo decreto-legge, nel riconoscere i diritti dei britannici in Italia. Abbiamo interesse a farlo, perché sono una frazione di quanti siamo noi nel Regno Unito, cioè sono meno di un decimo di quanti siamo noi; vogliamo vederci riconosciuti con reciprocità gli stessi diritti e quindi facciamo bene ad estenderli.

di alcuni argomenti con la questione Brexit, sulla quale congruità non entro, perché ovviamente è tutt'altro), abbiamo sottovalutato i i diritti e i bisogni dei cittadini italiani nel Regno Unito. Vi faccio notare che, su una ventina di articoli, ce n'è uno solo che riguarda i numerosissimi (700.000) cittadini italiani nel Regno Unito e concerne il fatto che c'è necessità di aumentare i servizi consolari a loro disposizione. abbiamo presentato una serie di emendamenti, che poi avremo modo di esporre e che tuttavia il Governo non ha ritenuto di accettare (e questo è grave), per specificare che queste risorse devono andare ai cittadini, quindi, se si assumono 50 funzionari consolari in più per la rete, questi funzionari devono andare nel Regno Unito. Nel Regno Unito c'è un funzionario consolare ogni 6.000 iscritti: 6.000 rispetto ai 330.000, quindi ce n'è uno ogni 12.000 effettivi, a fronte di uno ogni 90 in Italia, in un Comune, per l'erogazione degli stessi servizi. Se non scrivete che, dei 50 funzionari in più che verranno assunti, una quota si spera consistente deve andare nel Regno Unito, vi state semplicemente scordando dei cittadini italiani nel Regno Unito. Se non scrivete che qualche soldo in più a favore dei consolati deve servire per la riapertura del consolato

ecco, se non lo scrivete, vi scordate un pezzo importante, vi scordate di adempiere al vostro dovere, come Governo, di fornire i servizi a questa grandissima comunità: gli italiani residenti nel Regno Unito.

signor Presidente, non mi può impedire di ritenere che questo decreto Brexit e questo argomento rappresentino davvero una pietra miliare nel fallimento di questa unità europea. La fuoriuscita di uno dei Paesi fondanti ed essenziali dell'Europa, di uno dei Paesi più importanti del nostro continente credo non possa non essere riconosciuta come, appunto, il fallimento dell'Europa degli eurocrati, il fallimento dell'Europa dei burocrati, il fallimento di un'Europa che non appartiene ai popoli europei, ma che appartiene piuttosto ad altre consorterie.

c'è stato questo *referendum*, che ha fatto uscire un'importante nazione europea, e magari anche riflettere nell'ottica che non avvengano altre fuoriuscite, nell'ottica, cioè, che l'Europa dal 26 maggio in avanti possa rinforzarsi e non avere più Brexit, Italexit, Germanexit, ma possa avere piuttosto una nuova vitalità, nella luce e nello spirito di quei Trattati che proprio qui da Roma diedero il "la" a un'Europa che ben poco aveva da spartire con quella che purtroppo oggi abbiamo fronte. Nel merito, Fratelli d'Italia - lo diciamo chiaramente - è solidale con il popolo inglese, è solidale con l'Inghilterra, è solidale con un popolo che ha deciso, assumendosene la responsabilità, il rischio e le conseguenze, di uscire dall'unità europea.

favorivano alcuni Paesi piuttosto che altri e che non ha saputo dare pari opportunità ai Paesi membri dell'Unione europea. Ecco perché siamo solidali e comprendiamo il popolo inglese, anche se certamente non auspichiamo che altre nazioni siano costrette da questa Europa ad uscire. Perché ciò non accada, però, occorre - lo ribadiamo con forza e lo chiederemo nelle piazze e a tutti gli italiani un'Europa diversa da quella a trazione di centrosinistra, che ha caratterizzato gli ultimi anni della nostra vita politica comunitaria. Bruxelles, peraltro, sempre a proposito di Brexit, ha ostacolato l'accordo. Parliamoci chiaro: se il *deal* ad oggi non è stato concluso è perché qualcuno ha fatto di tutto affinché ciò non accadesse, perché si volevano ammonire i Paesi europei che dall'Europa, una volta entrati, non si può più uscire, magari come in certe consorterie più o meno legali, dalle quali, una volta che si è entrati, non è possibile uscire; quelle consorterie che tanto peso hanno in certi ambienti vicini agli eurocrati e ai burocrati di Bruxelles. Ebbene, se questo era il messaggio che voleva dare l'Europa, se è per questo che il *deal*, l'accordo consensuale, non è stato ancora trovato, ecco che doppiamente siamo solidali con il popolo inglese. Doppiamente Fratelli d'Italia si adopererà perché l'accordo non sia punitivo, ma sia rispettoso di un popolo, che aveva buone ragioni per dire no a questa Europa. D'altra parte, ricordo a me *in primis* e a noi tutti, che quello inglese è un popolo che non si è fatto spaventare da Napoleone e neppure da Hitler e certamente non si è fatto spaventare e non si spaventa per il signor Juncker o per i suoi collaboratori di Bruxelles e dell'Unione europea. Quindi, solidarietà piena e totale ad un popolo e ad una nazione che dovranno trovare un accordo bonario e costruttivo con l'Italia e con il resto dell'Europa. Brexit significa anche dare delle risposte al tema dell'immigrazione e a quelle politiche immigrazioniste che il Regno Unito non accettava e che invece hanno caratterizzato, come ho ampiamente detto ieri, la politica dell'Unione europea, a trazione di centrosinistra. La Brexit vuol dire anche un maggior rispetto, da oggi in avanti, per le patrie, per i territori e per la sovranità nazionale. Se vogliamo costruire davvero un'Europa dei popoli, dovremmo partire dal rispetto per i popoli nazionali dell'Europa, dal rispetto per le tradizioni e per le necessità dei territori europei. Quindi speriamo davvero che la Brexit significhi al più presto, possibilmente nei tempi autunnali previsti, un accordo non punitivo - lo ribadisco - che possa dare risposta

che questi nostri concittadini vengano tutelati, nel momento in cui non ci fosse un accordo per la fuoriuscita della Gran Bretagna. Dobbiamo tutelare le nostre esportazioni, il nostro *made in Italy*, i nostri prodotti ad indicazione geografica ad indicazione geografica tutelata e protetta. Dobbiamo avere riguardo alle comunicazioni, alle vie stradali e ferroviarie e ai nostri giovani, che tanto si sono resi protagonisti con i programmi Erasmus. Tutti questi aspetti vanno considerati nei rapporti con uno Stato europeo che se ne va da questa Unione europea.

però credo che se la maggioranza avesse avuto un atteggiamento costruttivo e, come ha detto prima un collega di Forza Italia, avesse saputo avere con le opposizioni un rapporto

in maniera forse quasi ossessiva, si concentra sugli aspetti tecnici di un passaggio estremamente delicato, quasi dovuto - anzi, direi dovuto - perdendo

in testa - spingeva per avere una grande area di libero scambio, con i Paesi dell'Europa dell'Est, che si affrancavano dall'influenza sovietica e potevano diventare interessanti dal punto di vista dell'*export* e dei servizi finanziari. Il Regno Unito insistette molto perché si andasse verso quel modello, che allargò certamente l'Unione e rese

meno. Un Paese come il nostro, che invece è stato tra i fondatori e ha spinto per un organismo sovranazionale straordinario, unico nel suo genere, uno sforzo di fantasia per affrontare le sfide del futuro, quelle che non si è in grado di affrontare con misure meramente nazionali; per sfide epocali come l'uscita dalle crisi economiche, la gestione dei flussi migratori, la lotta ai cambiamenti climatici, la lotta alla criminalità organizzata ci vogliono spalle larghe e una dimensione più ampia. Un Paese come il nostro, che è stato sempre nella prima fila degli Stati che hanno spinto per la costruzione europea, non può affrontare questo passaggio come se fosse meramente tecnico. È certamente giusto discutere su come mettere in sicurezza gli istituti assicurativi e bancari, le autorità di pagamento, su come rafforzare la presenza consolare e i servizi offerti agli italiani che risiedono nel Regno anche essere l'occasione per riflettere su cosa significhi questo passaggio per l'Europa. Vuol dire mettere in discussione i principi e i valori fondamentali che hanno fatto sì che questo fosse un esperimento straordinario: il tema dell'integrazione e della libera circolazione dei beni, dei servizi e delle persone, il fatto che ci si possa curare in tutti gli ospedali e le strutture sanitarie dei Paesi

senatore Comincini, collaborando con la Commissione, a porre ad esempio il tema di come, in assenza di norme chiare, si metteranno a rischio i voli con il Regno Unito, che uscirebbe dallo spazio comune, in cui ci sono regole condivise. Questo vale per tantissimi altri esempi che potremmo fare.

bilancia commerciale. Cosa succederebbe il giorno dopo? Varrebbe la clausola della nazione più favorita? Varrebbero le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio? Cosa facciamo noi per garantire e tutelare il sistema economico imprenditoriale?

(molti dei prodotti che esportiamo), il prodotto principe, ad esempio, ha il 35 per cento dei dazi. Se non si interviene anche da questo punto di vista, se non ci si muove in sede di Organizzazione mondiale del commercio, rischiamo di mettere in difficoltà una parte importante del nostro sistema economico e imprenditoriale. Questo vale anche per le barriere non tariffarie: molto spesso noi sottovalutiamo cosa significhi, perché ormai è entrato nel nostro modo di essere e di muoverci, nel nostro modo di fare impresa all'interno dell'Unione europea. Verrebbero inserite le barriere non tariffarie e questo vorrebbe dire le dogane; comporterebbe grandi ostacoli dal punto di vista burocratico per il nostro sistema imprenditoriale; questioni che non ci ponevamo più e che oggi, invece, ci troveremmo ad affrontare nuovamente. Tutto ciò vale anche per i cittadini italiani che si muovono per lavoro, per studio, vanno a studiare all'estero o fanno una breve esperienza professionale. È chiaro che per molti non sarà più possibile perché per circa 700.000 persone - un numero enorme - quello è il principale punto d'approdo: per i nostri giovani che vogliono andare all'estero, e non solo

nella capacità di muoversi dentro uno spazio unico europeo che garantisce queste libertà, lo possono fare. In futuro non sarà così perché ci vorranno regole molto più complicate per poter lavorare, per studiare, per andare a formarsi,

permessi di soggiorno e sul tema delle assenze, perché se siamo più aperti costringiamo, dentro un sistema di reciprocità, anche il *partner* del Regno Unito - in caso di non accordo - a dare questo tipo di garanzie. Concludo con un appello: questo non sia solo un provvedimento tecnico, ma sia affiancato da un dibattito e da una discussione seria perché la Brexit rischia di essere un *boomerang* per quei partiti e soggetti populisti che parlano di «prima i nostri». Alla fine, con questi tipi di politica, le promesse che fanno all'elettorato nel momento della campagna elettorale rischiano di ritorcersi proprio

Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, siamo qui a discutere del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 22 del 25 che reca misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea. Lo abbiamo detto a più riprese sia come maggioranza parlamentare che di Governo: l'Italia si farà trovare pronta in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Abbiamo mantenuto la promessa, e ringrazio per questo i membri del Governo coinvolti e i miei colleghi in Commissione per il prezioso lavoro svolto. La ricerca della stabilità, della tutela e della sicurezza degli interessi italiani rimangono per noi l'obiettivo centrale della nostra azione politica. Vado brevemente a illustrare i contenuti del provvedimento in esame, che introduce, come detto, misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati e ha l'obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale e della situazione relativa al Regno Unito. Il decreto-legge, in particolare, reca disposizioni che disciplinano diversi ambiti specifici, come ad esempio l'esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, misure dirette a disciplinare le conseguenze del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione europea e da ultimo, il mantenimento, con alcune necessarie modifiche, dello schema di concessione della garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze. Il provvedimento si componeva originariamente di 24 articoli, poi integrati da alcune modifiche inserite durante il lavoro di Commissione, che hanno apportato miglioramenti al testo in esame. Nella prima parte del provvedimento si trovano le disposizioni in materia di quei poteri speciali relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Vengono Vengono inseriti tra le attività di rilevanza strategica, e quindi soggette al *golden power* del Governo, i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati su tecnologia 5G. Una modifica importante, che tiene conto dell'evoluzione del contesto internazionale (ed ecco il perché dell'inserimento in questo decreto-legge) che tutela l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, riconoscendo l'importanza strategica di tale settore. Nella seconda parte del provvedimento vengono trattate una serie di misure volte a garantire la stabilità finanziaria. A riprova della lungimiranza del Governo, che ha scelto di arrivare preparato a un'ipotesi di *no deal*, un'intera sezione riguarda esclusivamente misure in caso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo. In particolare, tale sezione, reca norme in tema di prestazione dei servizi e delle attività in Italia da parte di soggetti del settore bancario del Regno Unito dopo la data di recesso, con particolare riguardo al periodo transitorio. Reca, inoltre, norme volte a garantire l'operatività dei gestori italiani di sedi di negoziazione del Regno Unito durante il periodo transitorio. Prevede inoltre disposizioni per la tutela dei depositanti e degli investitori, stabilendo che le banche del Regno Unito che alla data di recesso svolgono in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani. All'interno del provvedimento vengono previste, inoltre, disposizioni per la tutela dei cittadini italiani. Viene disposta l'equiparazione dei cittadini del Regno Unito ai cittadini dell'Unione europea ai fini della concessione della cittadinanza, in caso risiedano da almeno quattro anni in Italia. Vengono previsti, inoltre, diversi stanziamenti per il potenziamento dei servizi consolari nel Regno Unito, nonché ulteriori disposizioni per la tutela dei cittadini italiani ivi residenti. Nella terza parte il provvedimento mira a perseguire gli obiettivi del Governo sul tema della tutela e della protezione del sistema bancario, disciplinando l'estensione della garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze. Nell'avviarmi alla conclusione, vorrei effettuare un passaggio politico sulla vicenda Brexit. Il 23 giugno del 2016, tramite un *referendum* consultivo, i cittadini del Regno Unito hanno votato in maggioranza per l'uscita dall'Unione europea. Abbiamo assistito sin da subito a schiere di intellettuali che, insieme al sistema mediatico internazionale, hanno gridato allo scandalo, al popolo ignorante e privo dei mezzi necessari per comprendere dinamiche politiche così complicate, e hanno criticato la legittimità del voto. Nelle ultime settimane, si legge sempre più spesso, che queste future elezioni europee, alle quali parteciperà anche il Regno Unito, saranno un vero e proprio secondo *referendum*. In caso di sconfitta dei conservatori sarebbe chiaro e lampante il cambio di idea del popolo del Regno Unito sulla questione Brexit. A riprova di queste tesi che vogliono screditare il risultato del *referendum*, viene citato il mancato accordo tra i membri del Parlamento del Regno Unito sulle modalità di uscita dall'Unione. Lo voglio dire forte e chiaro: non è possibile dare adito a tali assurdità. Va chiarito, senza timore di smentita, l'incapacità manifesta della politica di tradurre in atti concreti le voci e i desideri dei cittadini, legittimamente espressi tramite un *referendum*. Non può diventare una scusa o un alibi per chi vuole a tutti i costi ribaltare il voto del giugno del 2016. La democrazia e la volontà popolare sono concetti sacri. Sono concetti che devono essere difesi sempre, non solo quando fanno comodo a qualcuno in particolare. Sono la base su cui si fondano le nostre democrazie ed è nostro dovere rispettarli. Con questo provvedimento noi dimostriamo di rispettare il popolo inglese e il processo della Brexit e adeguiamo il nostro ordinamento per tutelare e garantire la sicurezza economica dei nostri cittadini e delle nostre imprese.

È kafkiano tanto da essere quasi autolesionista: è scritto per un'ipotesi che non si realizzerà e riesce invece a realizzare benissimo alcune cose, cioè smascherare e rendere inefficaci alcuni presupposti politici sui quali si basava l'azione politica di questa maggioranza; parlo del fastidio enorme verso l'Unione europea, del fastidio verso i tecnici competenti e del fastidio verso il mondo della finanza. Questa maggioranza, molto infastidita dall'Unione europea, in questo caso cosa fa? Prende una comanda dall'Unione europea e scrive un decreto-legge in tre atti: nella prima parte, come hanno elencato benissimo le colleghe Tiraboschi e Modena che mi hanno preceduto, recepisce gli aggiustamenti previsti dall'Unione europea sulle Gacs, cioè sulle garanzie e sulla cartolarizzazione dei crediti; mette un cappio al collo sul mercato libero del 5G, creando addirittura questo gruppo di coordinamento che rallenterà moltissimo i rapporti commerciali e tutto quello che dovrebbe essere fluido, negando anche la possibilità del Parlamento di essere informato (quindi, davvero un capolavoro); infine scrive, facendosi aiutare dai tecnici, un provvedimento che non si realizzerà mai, perché sappiamo che il decreto Brexit si applicherà solo nel caso di *no deal*. Adesso c'è stata una proroga fino ad ottobre, e un *deal* in qualche maniera ci sarà sicuramente. La seconda questione politica è che questa maggioranza, talmente incattivita con i tecnici, si è fatta proprio scrivere tutti gli articoli del decreto Brexit dai tecnici. Noi li abbiamo auditi in Commissione finanze: abbiamo audito il MEF, la Banca d'Italia, la Consob, La maggioranza, interrogata da una minoranza incalzante che voleva essere sicura che dal punto di vista economico-finanziario ci fosse tutto quello che dovesse esserci per scongiurare ogni tipo di buco normativo, ha detto: «sì, sì, certamente: se n'è occupato il tavolo tecnico del Fantastico, questa è una notizia politica: ora noi tutti sappiamo che la maggioranza ha stima e si fida dei tecnici. Noi che, da meritocratici, dei tecnici competenti ci siamo sempre fidati e abbiamo sempre collaborato in maniera proficua, ai tecnici però chiediamo una cosa, visto che gli interlocutori di questo decreto-legge sono loro: come mai non hanno modificato gli articoli 3 e 4 del decreto-legge? Faccio riferimento in questo caso ai servizi di investimento, perché forse si sono un po' confusi ed è rimasta una lacuna nella norma. Qui è previsto solo che i servizi di investimento vengano svolti dalle banche. In realtà non sono svolti solo dalle banche, ma anche dagli intermediari finanziari, dalle SGR, dagli OICR, dai gestori dei mercati regolamentati. Se quindi, nel frattempo che scrivono gli ultimi emendamenti, correggono e recepiscono anche questo utile suggerimento, magari dal punto di vista tecnico il decreto-legge risulterà perfetto, come naturalmente i tecnici l'hanno scritto. la cosa veramente incredibile è che questa maggioranza, che ha fatto una campagna elettorale per i precedenti cinque anni contro le banche e contro il mercato della finanza, ha scritto, approvato ed è

invece hanno una ricaduta reale sui popoli, sulla vivibilità di questa Unione europea. Si tratta di una lacuna talmente grave che si è meritata un richiamo scritto e formale, che abbiamo letto in 6a Commissione questa mattina, da parte della Presidente del Senato, che giustamente ha fatto notare che il decreto-legge, dal punto di

questa maggioranza con questo decreto-legge di fatto non ha compiuto passi avanti perché non si applicherà mai. Ha però fatto un'enorme operazione di verità dicendo che sta rinnegando tutti i presupposti politici per i quali i cittadini li hanno votati. Ebbene questa è una notizia. una seconda notizia altrettanto importante: questo decreto-legge è autolesionista. È pur vero che è stato scritto dai tecnici parlando di banche, di mercati e di finanza, però di fatto giustamente - perché i tecnici lo scrivono così - non si occupa degli interessi reali della finanza e dei mercati. Non se ne occupa perché questo è un decreto-legge di "divorzio"; è un decreto-legge che regola le fattispecie di divorzio tra il Regno Unito e i Paesi dell'Unione europea e, in questo caso, l'Italia. Dal Dal punto di vista strategico-politico, forse l'unico suggerimento che la maggioranza avrebbe dovuto dare è come regolare le fattispecie affinché gli operatori che operano in Italia possano continuare a farlo in ogni caso. Non stiamo Non stiamo parlando proprio di nulla: stiamo parlando di 70 banche britanniche, 223 istituti di pagamento, 100 emittenti di moneta elettronica, 21 fondi (che assicurano poi il 12 per cento delle prestazioni previdenziali) e 58 compagnie assicurative. Stiamo parlando dei cardini dei rapporti economico-finanziari bilaterali tra Italia e

è che è stata un'esercitazione che però vi è riuscita male e anche in termini pericolosi. Noi, infatti, in Commissione finanze abbiamo visto

europei, l'Italia è tra i meno esposti con l'Inghilterra, sia sul piano commerciale che sugli investimenti, pesando il Regno Unito sugli scambi di beni poco più del 5 per cento sull'*export* italiano, contro il 7 per cento di Francia e Germania, e oltre il 10 di Paesi Bassi e Irlanda. Tuttavia l'Italia, avendo un consistente *surplus* commerciale con il Regno Unito - oltre 10 miliardi di euro l'anno - in costante aumento, con la Brexit subirebbe un impatto importante sull'economia, in particolare su alcuni settori di punta del nostro *export*, come la meccanica strumentale, il tessile, il chimico e l'agroalimentare. Per garantire stabilità finanziaria e integrità dei mercati, tutelare investitori e clientela, il decreto-legge prevede un regime transitorio differenziato in base alla natura dei soggetti e del tipo di attività. Alle banche, alle imprese di investimento e alle succursali italiane degli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito viene concessa la possibilità di continuare a operare per altri

queste banche ed imprese di investimento abilitate a partecipare alle aste di titoli di Stato non è richiesta la presentazione della notifica, salvo che per continuare a esercitare la raccolta del risparmio. In tal caso, dopo aver presentato l'istanza di autorizzazione, gli intermediari potranno continuare a esercitare l'attività per diciotto mesi dalla data di recesso. Per le banche che operano in modalità di prestazione di servizi senza stabilimento viene prevista una limitazione alla raccolta del risparmio consentita solo per i rapporti esistenti - in attesa dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione a operare come banche di Paese terzo. Le attività svolte da tali soggetti sono sottoposte alla normativa bancaria e finanziaria europea e nazionale, inclusa quella in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, usura, trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. Il riconoscimento per banche e imprese di investimento del Regno Unito a proseguire la propria operatività vale anche per l'abilitazione alle aste di titoli di Stato e per la qualifica di specialista in titoli di Stato e dei profili di partecipazione alle infrastrutture di *post*-*trading*. La possibilità di continuare a prestare servizi di investimento - nei limiti previsti dalle disposizioni transitorie - consente di gestire le potenziali ricadute connesse a un *no deal* per il servizio dei contratti derivati *over the counter* (OTC) conclusi da intermediari del Regno Unito con soggetti italiani. Tali intermediari, ai quali non è consentito di assumere lo *status* di intermediario di Paese extra-UE e quindi di poter operare in Italia con succursale o in regime di prestazione senza stabilimento, dovranno procedere in sei mesi alla cessazione delle attività o alla cessione dei rapporti a soggetti autorizzati. A tutela dei risparmiatori, per i finanziamenti concessi la cessazione del rapporto non modifica i termini e le modalità di pagamento degli interessi e del rimborso del capitale. Si introduce un regime speciale per la gestione dei contratti derivati contratti derivati OTC in essere tra controparti italiane e imprese di investimento del Regno Unito che non intendano richiedere l'autorizzazione ad operare in Italia o a cedere i rapporti instaurati a un intermediario italiano. In tema di continuità contrattuale, la Commissione europea ha approvato modifiche ai regolamenti delegati relativi all'obbligo di *clearing* e allo scambio di garanzie su base bilaterale per i derivati OTC, che incoraggiano la sostituzione - tramite la novazione - delle controparti dei contratti OTC del Regno Unito con controparti stabilite nell'Unione, prevedendo una finestra di dodici mesi, a decorrere dalla data della Brexit. Il decreto-legge prevede specifiche disposizioni anche per il settore assicurativo a tutela degli assicurati, per consentire alle imprese del Regno Unito, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge siano già abilitate ad operare nel territorio della Repubblica, di proseguire l'attività limitatamente alla sola gestione dei contratti e delle coperture in essere, fino al diciottesimo mese successivo all'inizio della Brexit. Per garantire la continuità dei servizi e prevenire ricadute sfavorevoli agli assicurati nel periodo di transizione le imprese dovranno procedere alla sola gestione dei contratti: non potranno stipulare nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, i contratti esistenti, poiché mancano i requisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano richiesti dalla normativa a causa del mutato quadro giuridico di riferimento. il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 è stato autorizzato, a seguito della decisione della Commissione europea, uno schema per la concessione della garanzia di Stato sulla cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, non qualificata come aiuto di Stato, con l'obiettivo di consentire l'avvio di un mercato secondario concorrenziale per la cessione di tali crediti deteriorati. Si tratta di un capitolo doloroso per le banche italiane e per i cittadini, con la valutazione data a seguito della direttiva BRRD e del *bail-in* che ha portato alle risoluzioni bancarie del 21 novembre 2015, mettendo in mezzo ad una strada 130.000 famiglie, pari al 17,6 per cento (questa è la valutazione). L'affare del secolo per fondi avvoltoi ed altri intermediari che lucrano fiorenti profitti sulla pelle dei cittadini, i quali, se espropriati, non possono neppure concorrere a riacquistare i beni cartolarizzati, il cui tasso di recupero per le banche è superiore al 45 per cento, contro un 26 per cento delle società veicolo. veicolo. In conclusione, signor Presidente e colleghi, da questa gabbia europea fondata sull'euro, una moneta senza popolo costata 73.605 euro ad ogni italiano e 4.325 miliardi di euro di mancata crescita negli ultimi venti anni (non lo diciamo noi ma il rapporto di una fondazione tedesca), è difficile uscire persino per chi aveva mantenuto la sterlina come segno monetario identitario. Ma, come già accaduto con il *referendum* in Grecia, la sovranità non appartiene più ai popoli ma alle consorterie finanziarie che decidono e continuano a decidere sui destini del mondo alla cui asfissiante egemonia cerchiamo di resistere evocando l'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo, non alle oligarchie. *(Applausi

Quindi, quando la senatrice si riferisce ai risparmiatori, vorrei dirle che questi prodotti che verranno fuori e che verranno costruiti dalle società veicolo di fatto non sono prodotti per risparmiatori ma per gli investitori, cioè per una figura diversa da quella del risparmiatore. Sono prodotti che saranno appetibili per le società di gestione del risparmio,

Per lo stesso principio, vorrei rispondere alla senatrice Conzatti quando fa riferimento all'articolo 3 del decreto-legge, lamentandosi del fatto che tale articolo preveda la possibilità, per le banche che ne fanno richiesta alla Banca d'Italia, di poter continuare ad operare con la clientela mentre la stessa previsione non è fatta nei confronti dei gestori di fondi e degli OICR.

la clientela istituzionale, la clientela professionale (privata e pubblica) e la clientela al dettaglio. Gli OICR, così come le società di gestione del risparmio, possono direttamente collocare i prodotti e avere rapporti con la clientela professionale, ma non con la clientela al dettaglio: con la clientela al dettaglio, possono farlo solo ed esclusivamente tramite le banche. Quindi, colui il quale abbia, per esempio, 500.000 euro di risparmi può direttamente avere rapporti con l'OICR o con la società di gestione del risparmio, ma anche fuori dell'Unione europea. Quindi, nel caso in cui il Regno Unito dovesse uscire, le società di gestione di risparmio e gli OICR del Regno Unito comunque potranno continuare ad avere rapporti con la clientela italiana, ma non con la clientela al dettaglio, perché della clientela al dettaglio se ne occupano esclusivamente le banche. Un'ultima osservazione vorrei poi farla nei confronti di coloro che esprimevano grande preoccupazione per l'eventualità che non fosse rispettato, nel decreto Brexit, il principio di reciprocità.

dovesse uscire dall'Unione europea, di tutelare le nostre imprese per quanto riguarda, per esempio, le esportazioni. Quindi, una tutela negli accordi bilaterali. Per quanto riguarda, invece, gli accordi in essere, non dimentichiamo che il popolo inglese è, probabilmente, per storia, tra i più democratici del mondo. Senatore Fantetti, lei su questo mi può dare Non dimentichiamo che il popolo inglese è quello che ha avuto la Magna Charta nel 1215 ed è stato l'unico popolo che ha avuto la capacità,

ma concludo, ringraziando il Governo al quale do fiducia. Sono convinto che riuscirà a gestire bene i rapporti bilaterali

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre 18 mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea ''*point to point*'', mediante aeromobili del tipo ''*narrow body*'' (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.».

Signor Presidente, per le condizione date ritengo che la formulazione proposta dal relatore sia quella che possa consentire di limitare, in questa fase, i possibili danni e le possibili criticità che l'operazione della Brexit può comportare all'aeroporto di Linate e più in generale al sistema aeroportuale lombardo. Auspico possa esserci in uno dei prossimi provvedimenti del Governo

2020, ma anche nel periodo futuro. Quindi, vigilerò perché anche questo possa avvenire e coopererò con la maggioranza e il Governo affinché si possa trovare la soluzione migliore.

Alla lettera *b)* scriviamo «valore del prestito al lordo delle rettifiche di valore (*gross book value*) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale titoli emessi».

Presidente, possiamo anche accogliere la richiesta del Presidente del Gruppo PD di accorciare i tempi e concludere

Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di un provvedimento che giustamente punta a tutelare gli interessi degli italiani e delle aziende italiane che vivono in Gran Bretagna. Non è nostro compito entrare nel dibattito e nelle decisioni che prenderà un altro Paese; tuttavia, alcune riflessioni sono necessarie. Concordo con ciò che ha detto in discussione generale il collega Fantetti per quanto riguarda l'entrata

quando si trattava di integrare di più l'Europa era sempre l'Inghilterra ad essere un freno forte. Bisogna conoscere questa storia per

oramai siano forti le relazioni all'interno dell'Unione europea; quanto siano consolidati gli scambi, la presenza di cittadini e imprese di uno Stato nell'altro.

si fa più caso. Siamo uno spazio unico, per cui l'unica strada possibile è quella di migliorarlo e non di distruggerlo. Non è vero che le istituzioni europee sono state troppo presenti, privando di sovranità gli Stati nazionali. Il problema è che, da un lato, gli Stati nazionali sono stati un ostacolo per dare uniformità istituzionale e politica a quanto nella società e nell'economia esiste già; dall'altro, l'Europa si è data un'agenda sbagliata, inseguendo tematiche e imponendo regole che sono apparse incomprensibili agli occhi dei suoi cittadini. Come Gruppo per le Autonomie chiediamo una nuova Europa, più forte e veramente unita: un'Europa che metta da parte gli egoismi e che giochi un ruolo da protagonista nel mondo. Un'Europa che è la somma di tante minoranze e dove tutti sono rispettati e protetti, dove si è fieri della diversità e della propria specificità, perché tutte le grandi democrazie nascono e crescono solo su queste basi. La demografia, prima ancora dei dati economici, ci dice che ogni Stato europeo non avrebbe nel mondo alcuna possibilità di contare qualcosa. Solo con l'Europa unita, solo con un Continente di 500 milioni di persone, le nostre comunità possono aspirare ad avere un ruolo rispetto ai grandi temi del futuro: il tema dell'ambiente e della sostenibilità ambientale del Pianeta; quello della sicurezza, che ogni giorno di più si intende come *cyber security*; quello della nuova rivoluzione industriale, con la piena automazione dei processi produttivi. Il sovranismo, come dimostra la vicenda inglese, non tutela un popolo, ma produce danni per gli uni e per gli altri: un danno perché quando più elementi si sono fusi è quasi impossibile poterli separare senza traumi. La vicenda di quel *referendum* dice moltissimo sulla cautela con cui vanno usati gli strumenti di democrazia diretta. Il *referendum* è una scelta netta, è l'impossibilità di ricomporre un quadro, è la fine di ogni possibilità di confronto e di mediazione. produce decisioni che non tengono conto delle conseguenze, soprattutto quando una delle due scelte non è reale, ma è solo l'avvio di un percorso inesplorato e pieno di incognite. In conclusione, Presidente, il nostro auspicio è che la Brexit possa essere da monito per tutti i cittadini europei e anche per quelli italiani. Spero che l'Italia riscopra la sua centralità in Europa. Un'Europa diversa, più forte e coesa non ci può essere senza la centralità di un Paese fondatore, della terza economia del Continente, di un soggetto determinante nei grandi passaggi per l'unificazione europea. L'Italia riscopra questo suo ruolo e si metta al centro del progetto per una nuova Europa. È con questo auspicio che rinnovo il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento.

il decreto-legge è una specie di atto dovuto in caso di *no deal*. Tutti auspichiamo al 31 ottobre

che se avesse avuto nella coalizione la maggioranza assoluta avrebbe indetto il *referendum* per confermare la presenza del Regno Unito all'interno dell'Unione europea. Il tutto sull'onda di di un percorso che fino ad allora era stato un crescendo tra le forze che auspicavano fortemente l'uscita

stavano incidendo fortemente nel tessuto più fragile. Noi pensiamo tutti a Londra, dove non ha vinto il *referendum* pro-Brexit, ma

ieri nel Parlamento europeo ha richiamato l'Unione europea e il Parlamento stesso a responsabilità più forti verso la transizione energetica e contro i cambiamenti climatici. La nuova Europa si deve fondare strettamente

sociali, fuori dal benessere di una grande capitale finanziaria come Londra, sono stati percepiti come il frutto

commerciali verrebbero regolati dalle norme del WTO e, per il primissimo periodo e il medio termine, sul *made in Italy* questo avrebbe un impatto fortissimo. Ma pensiamo anche all'impatto sui viaggiatori, sui consumatori, sugli studenti, sui residenti. Noi abbiamo tra i

hanno fatto sì che ci fosse una condivisione più ampia. Per tutti questi motivi riconfermo il nostro voto favorevole.

inconsapevolmente, almeno per quanto riguarda forse le aspettative del Governo, racchiude in sé quanto sta cambiando nella politica europea, nella politica internazionale e il problema del nostro Paese. Lo racchiude nel titolo, che riguarda giustamente misure urgenti per garantire sicurezza, stabilità finanziaria, integrità dei mercati, e soprattutto per tutelare i nostri cittadini e le nostre aziende in Gran Bretagna dopo l'uscita che verosimilmente ci sarà (quando ci sarà, lo vedremo). Ma lo racchiude anche perché inconsapevolmente il Governo, pensando di utilizzare come veicolo questo decreto-legge, ha inserito l'altra grande frontiera della politica internazionale del nostro Paese,

bloccare, attività ostili nei nostri confronti per il controllo del sistema Paese che, attraverso la tecnologia 5G, chiunque può realizzare

sui dati e, quindi, sull'economia della conoscenza, che oggi sostanzialmente presiede e pervade di sé ogni forma economica, politica e sociale (come dimostrano i casi di democrazia diretta e anche di incursione elettorale), l'avremmo voluta estendere a tutto ciò che riguarda il settore della banda larga. Nel contempo - lo dico ai colleghi parlamentari

che le consente di tutelare in modo specifico tutta la tecnologia utilizzata dai servizi di sicurezza, di tutela e di difesa della propria Nazione. Queste sono le nostre due direttrici emendative che non so se consapevolmente o inconsapevolmente - la maggioranza ha respinto. Davamo al Governo e al Ministro dell'interno la facoltà di poter tutelare meglio la sicurezza nazionale anche per quanto riguarda l'aspetto della tecnologia, proprio utilizzando la normativa francese, che su questo è molto più pregnante della nostra. Purtroppo, non è stato possibile perché forse a questa maggioranza

della nostra Unione europea, che aveva preso le mosse in Italia con i Trattati di Roma sulla base di tre Nazioni che all'epoca avevano la stessa dimensione demografica, economica

insieme ai tre Paesi più piccoli, cosiddetti cuscinetto, e cioè i Paesi del Benelux. L'architrave iniziale dell'Europa poggiava su tre Nazioni paritetiche. Poi, l'ingresso della Gran Bretagna in qualche misura, ci ha aiutato perché era una quarta nazione su cui noi spesso ci appoggiavamo per evitare che l'asse europeo fosse sbilanciato dalla riunificazione tedesca, cioè dalla calamita tedesca a cui spesso i francesi si assoggettano. Per tanti anni - chi ha fatto politica nel Consiglio europeo lo sa bene - noi appoggiati alla Gran Bretagna e la Gran Bretagna si è appoggiata all'Italia (penso soltanto alla politica occidentale di Berlusconi, con Blair e con Aznar, al di là della collocazione dei Governi e della politica atlantica di quelle nazioni). Questo riequilibrio, determinato

dove si è formato questo nuovo asse di Aquisgrana. Le elezioni europee tra pochi giorni ci consentiranno forse di imboccare un'altra direttrice, ma è assolutamente necessario che lo faccia l'Italia, perché è l'unico Paese escluso può rimettere in moto un equilibrio paritetico tra le nazioni europee, una nuova architrave con un nuovo progetto. Penso che per tale motivo questo decreto-legge, contenendo inconsapevolmente sia la minaccia cinese (cioè la nuova frontiera d'Oriente che entra in Europa) che l'uscita dalla Gran Bretagna, ci impone di riflettere su quale sarà il ruolo dell'Italia nei prossimi anni e quale sarà - se ci sarà - il futuro del nostro Paese in Europa. Presidente, siamo arrivati al lavoro in Aula dopo un importante lavoro istruttorio in Commissione,

in ragione del fatto che il provvedimento ha un valore ordinamentale e siamo passati da circa 90 proposte di emendamenti a 50 votazioni riferite a emendamenti ritenuti idonei dal punto di vista dell'istruttoria.

Una prima verità emerge: non è detto che ogni volta, per conoscere, per appurare e diventare consapevoli ci sia bisogno di sbattere il muso

determina poi una presa di coscienza che nasce purtroppo dalla durezza della realtà. Vi ricordate i mesi del 2016,

Ogni realtà territoriale provava a configurarsi con la categoria dell'Exit. Ho potuto leggere su una importante rivista internazionale che si arrivò a teorizzare addirittura di una nuova maniera di essere moderni: l'importante era allontanarsi, discostarsi, mettere in discussione. Abbiamo adesso rilevato come non è vero che il male assoluto è l'Europa ma si tratta di coniugare una nuova lettura di ciò che dall'Europa ci dobbiamo attendere. Mettiamo in discussione la qualità e la quantità della cittadinanza europea, quanto ci deve dare in più, su cosa porta in più rispetto alla cittadinanza nazionale, o tutta la partita delle infrastrutture che devono assicurare più qualità nei trasporti, o anche immaginare, per esempio, rispetto all'Europa, la configurazione di una sicurezza internazionale

la capacità di continuare a vivere e operare di persone, imprese e infrastrutture; persone nella loro diversa declinazione: quando studiano, quando investono, quando si curano, quando vogliono realizzare un progetto di vita. Anche per le infrastrutture della connessione aerea abbiamo fatto in modo che la dicitura di nazionalità non determini poi difficoltà di connessione internazionale con il nuovo stato terzo che è l'Unione europea nei confronti della Gran Bretagna. Noi avremo una nuova configurazione giuridica

modo abbiamo discusso di infrastrutture digitali relative alle informazioni che devono velocizzarsi attraverso il 5G senza perdere sicurezza, sovranità e integrità nazionale. Su questo abbiamo lavorato rispetto all'articolo 1 facendo in modo che i progetti di investimento tecnologico e digitale del 5G abbiano, sì, l'informativa e l'autorizzazione di Palazzo Chigi, ma abbiamo anche concordato la presentazione, a breve, di un decreto del Presidente del Consiglio per far sì che i tempi di istruttoria siano stabiliti, per evitare che si allontanino gli investitori. La lezione che arriva da questo da questo decreto-legge è una lezione - permettetemi - di moralità politica riferita a coloro i quali non volevano mai trovarsi a l'eterogenesi dei fini. È straordinario che un Governo sovranista, nazionalista abbia dovuto trovare una soluzione con un decreto-legge riferito proprio al superamento, all'allontanamento, all'uscita dall'Europa. Nei fatti, oggi abbiamo ricentrato il rapporto tra il sistema delle realtà nazionali e l'Europa. Ciò comporta una lezione e ci fa dire che dobbiamo mettere al riparo gli elementi costituzionali, istituzionali e ordinamentali rispetto al dibattito ideologico, che infanga la ragione e che fa in modo che tutto venga ammatassato salvo poi essere costretti a trovare rimedio. Abbiamo lavorato

Sul piano dell'istruttoria e anche del merito, abbiamo lavorato per fare in modo, per esempio, che gli aeroporti del sistema Italia, ma non solo, non venissero bloccati da Brexit perché non è giusto

che aveva fertilizzato come la via d'uscita da ogni problema l'ipotesi della Brexit. È su questo che parte, significativamente, un incasso, una patrimonializzazione della classe dirigente italiana e della comunità nazionale italiana. Evitiamo di ridurre tutto ad una specie di confronto tra tifoserie. Cerchiamo di coltivare il merito, approfondendo ciò che succede dopo. Se si fa questo, che succede dopo? Noi abbiamo appreso, per esempio, che la domanda etica

per i cittadini, per le imprese, per la capacità del sistema economico di essere competitivo oppure sdraiamo tutto a terra e gettiamo il Paese in quella incertezza che c'è adesso in Gran Bretagna? Provate a stimare chi, adesso, in Europa prova ancora a sorridere adesivamente rispetto alla scenata dell'uscita dall'Europa. Invece, la partita è discutere nel merito, configurare meglio, precisare, cercare, insomma, che, da un quadro di cooperazione, vengano più diritti, più certezze, più funzionalità e non l'ossequio ad una ideologia impazzita, che già in questa sede ci ha fatto misurare l'errore. Per questo motivo, noi votiamo a favore rispetto al decreto Brexit convertito in legge.

una materia - vorrei dire - inutilmente complessa. Forse, dovremmo anche interrogarci sul perché la matassa da districare fosse così complicata. Vorrei partire dalle tante interessanti sollecitazioni che sono arrivate nelle dichiarazioni di voto precedenti, per chiarire che non vi è alcun paradosso se una maggioranza, che si è posta come principio di azione politica la tutela dell'interesse nazionale, interviene per tutelare l'interesse nazionale a condizioni di reciprocità. Viceversa, quello che ci sembra un po' paradossale, e da cui dobbiamo trarre lezioni, è, probabilmente, l'atteggiamento di quella che io, non per pedanteria, ma per quel minimo di chiarezza che occorre in una sede come questa, continuo a chiamare Unione europea. Quindi, io parlo di progetto unionista e non di progetto europeo. L'Europa è un'altra cosa: c'era prima di noi, c'era prima dell'Unione europea, ci sarà dopo di noi e ci sarà dopo l'Unione europea, che è solo uno dei modi che abbiamo scelto per organizzarci politicamente; forse, non il modo più efficiente. Io vorrei ricordare, tanto per chiarire da che parte stia l'ideologia impazzita, una simpatica dichiarazione del 20 maggio 2016, che ancora trovate sul sito della Reuters, quando Jean Claude Juncker si espresse così: «i disertori britannici non avranno alcuno sconto dall'Unione europea». Dei toni così bellicosi, da parte di un progetto che viene ancora visto, dalla minoranza di questo Parlamento, come irenico e come responsabile dei famosi settanta anni di pace (che in in verità ci ha dato la Nato) sono quantomeno incongrui. Questo atteggiamento di minaccia ha creato una situazione abbastanza strana. le cose sono andate come dovevano andare, è stato chiaro che il progetto unionista si trovava ad un bivio e aveva di fronte a sé due strade ugualmente sbagliate. il progetto unionista poteva: o rispettare la scelta dei cittadini britannici, che stavano semplicemente esercitando un diritto garantito loro dai Trattati, e che, quindi, non meritavano per questo di essere minacciati dalle massime autorità europee, che di quei Trattati erano i difensori,

si rivelava una cosa evidente, cioè che questo progetto non era così attraente come lo si voleva proporre. *(Applausi dai Dall'altra parte, andando avanti con la minaccia (questa è la strada che si è scelta) si è fatto un danno ancora peggiore, perché si sono creati dei costi di transizione inutili: noi siamo stati qui a districare tutta una matassa

negoziatore Barnier ha fatto sua la filosofia di chi lo ha messo lì, il signor Selmayr, arrivato alla posizione di rilievo che occupa attraverso un procedimento sul quale ci dovremmo tutti interpellare e su cui l'*ombudsman* della Commissione europea ha espresso tanti dubbi,

voler punire il Regno Unito si è già rivelato, da parte di chi c'è dietro a questo negoziatore, cioè da parte della potenza egemone, la Germania, un errore piuttosto grave. In questo In questo strano *game of chicken,* come nella scena del film «Gioventù bruciata», invece che James Dean abbiamo Barnier al volante, ma non glielo abbiamo dato noi; sulla macchina ci siamo noi e la gioventù bruciata sono i nostri figli, il cui futuro è messo a rischio da questo modo spregiudicato

da questo episodio della storia europea; dobbiamo realmente tener conto del dato di fatto che purtroppo l'Unione europea si rivela una volta di più un luogo particolarmente inefficiente di mediazione degli interessi nazionali, degli interessi di comunità che si raccolgono sotto una Costituzione all'interno di uno Stato, rappresentate da Parlamenti democraticamente eletti. La mediazione europea è particolarmente inefficiente e trasforma un gioco un gioco a somma nulla in un gioco a somma negativa. Questo mi sento di dire. Dall'altra parte basta vedere cosa succede. Noi siamo qui con il paradosso di un sistema al quale chiediamo di assicurare prosperità e pace, che piange il lutto di un mercato finanziario, quello di Londra, che se ne va dimostrando così di non essere capace, non solo di creare politica, ma neanche di creare un mercato. Siamo qui di fronte al paradosso di persone di intonazione liberale che piangono il lutto di un monopolio, quello del mercato borsistico di Londra; quindi l'aggressione da parte dell'Europa (in particolare della Germania) al Regno Unito è qualcosa che rivela la profonda irrazionalità (per la quale noi naturalmente amiamo i nostri fratelli tedeschi, ma che spesso li ha caratterizzati), il loro profondo idealismo e la loro totale assenza di pragmatismo. Non dimentichiamo infatti che il Regno Unito è cliente della Germania e non si è mai visto nel mondo un commerciante che prendesse a calci nel sedere o che minacciasse un suo cliente. Questo è lo spettacolo che ci danno i nostri fratelli tedeschi, con i quali allearsi qualche nostra storia, di tanto in tanto, si è rivelato un errore. Allora, a fronte di tanta irrazionalità e incapacità di gestire per il bene della comunità europea un processo che i Trattati comunque disciplinavano e prevedevano, è chiaro che non ci può essere altro che uno sguardo di profonda attenzione critica verso

riflettere seriamente e serenamente su come gestire la situazione nella quale ci siamo venuti a trovare. In questa particolare contingenza il Governo italiano ha affrontato con senso di responsabilità

eventualmente per accadere, cioè l'uscita di un Paese dall'Unione europea, la minaccia non è tanto nella scelta di chi l'ha compiuta, quanto nell'atteggiamento di chi, dall'altra parte, non l'ha accompagnata, ma l'ha gestita con spirito di contrapposizione, per dare una punizione esemplare che, come metodo politico, ritenevamo e speravamo appartenesse ad epoche che pensavamo di esserci lasciati alle spalle. *(Applausi

Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori del Governo, il provvedimento oggi in esame prevede le disposizioni che dovrebbero essere adottate in ipotesi di uscita del Regno di Gran Bretagna dall'Unione europea, senza che si raggiunga alcun accordo (cosiddetto *no deal*). Una breve premessa: il Governo inglese ha richiesto e ottenuto più rinvii per la sua decisione. Giorni fa i Capi di Stato dell'Unione europea hanno proposto una ulteriore possibile proroga della decisione, addirittura al 31 ottobre prossimo venturo, ponendo però, a mio avviso, rilevanti problemi al funzionamento delle istituzioni europee, date anche la concomitanza delle elezioni del Parlamento previste per il periodo dal 23 al 26 maggio. A tale proposito, rammento che la signora May ha dichiarato l'8 aprile che, in caso di voto favorevole del suo Parlamento all'uscita con accordo, tale evento, avverrà in data 22 maggio e quindi il Regno Unito non parteciperà alle elezioni europee. A chi scrive sembra che questo continuo rinvio si atteggi a una vera e propria farsa: farsa: chi dice "restiamo", chi dice "usciamo", chi paventa problemi di ordine pubblico, chi addirittura fa previsioni catastrofiche di decisioni per l'autonomia da parte dell'Irlanda un vero caos. ha affermato che sotto il profilo economico la sua nazione, in uscita senza accordo, subirebbe un aumento di almeno il 15 per cento per i generi alimentari e dell'8 per cento per quelli tessili; un vero danno per i consumi del ceto medio-basso. Aggiungasi inoltre che il Regno Unito, ulteriore posta negativa, dovrà versare all'Unione europea ben 40 miliardi di euro, in gran parte nel periodo dal 2019 al 2025. Non entrerò nel merito del provvedimento, composto di 24 articoli, già chiaramente illustrati da coloro che mi hanno preceduto. Rammento solo che le disposizioni, che mi auguro non entrino mai in vigore, tendono a tutelare gli istituti bancari ed assimilati di entrambe le nazioni, sempre ovviamente in ipotesi di recesso, le prestazioni di servizi in Italia e in Gran Bretagna da parte sia dei soggetti italiani che di quelli inglesi, la tutela, anche fiscale, dei cittadini delle due nazioni e le regole per la loro permanenza nelle due nazioni anche in ipotesi di soggetti non cittadini, ma di lunga residenza. Viene infine prevista - fatto questo di rilevanza non indifferente la sostituzione del capitale versato dalla Gran Bretagna nella Banca europea degli investimenti, con l'accollo di tale onere, *pro quota*, agli Stati membri. Altro elemento negativo è quello che, sempre in ipotesi *no deal*, comporterà, sia per i cittadini sia per gli imprenditori, una serie di iniziative non sempre semplici e gradevoli, dovendosi recare forse più e più volte presso le rispettive ambasciate o uffici consolari, al fine di regolarizzare la propria permanenza o attività nei rispettivi Paesi. Un ulteriore effetto negativo si avrà, quasi sicuramente, per l'economia nazionale, in quanto verranno imposti, per le importazioni nel Regno Unito, dazi e altri balzelli anche burocratici,

rilevanza, essendo solo il 5 per cento del totale. Sulla base di tutti questi argomenti, confermando l'augurio che si vada ad un'uscita del Regno Unito con apposito accordo, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia.

le osservazioni approfondite e ispirate che sono state fino ad ora avanzate, per tentare, se possibile, una sintesi del dibattito odierno,

soggetti che, in qualche modo, esprimono una sorta di ribellione rispetto a questa Europa, ma mi chiedo quanto di questo sia genuino e spontaneo

Certamente il titolo del provvedimento in esame non è ottimistico, perché parla di un'Europa del futuro o del futuro di un'Europa nel cui contesto non ci sarà più il Regno Unito.

Invece, ci dobbiamo occupare di questioni economiche. È l'economia che corre al passo con la politica; è la politica che talvolta, come in questo caso, non riesce nemmeno a gestire i fatti economici. Per questo siamo qui con il provvedimento in esame. Non intendo soffermarmi sui contenuti tecnici del decreto-legge in oggetto, perché sono stati già ampiamente dibattuti e - comunque - questo è un provvedimento necessario e opportuno per mettere in sicurezza i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei nostri cittadini, consumatori e aziende. È con orgoglio che rivendico come l'Italia sia arrivata tra i primi Paesi a difendere giuridicamente gli interessi dei propri cittadini davanti

L'Europa che resta, ha sufficientemente riflettuto sulle ragioni che hanno spinto il popolo inglese a decidere così come ha fatto?

In realtà, quello che è accaduto, signori, è che abbiamo assistito all'epilogo di un processo di sfiducia che ha colpito una parte della cittadinanza europea fino al punto che questa non è più riuscita a intravedere una prospettiva di crescita. Quello che è successo in Inghilterra è una sorta di condizione di malessere che ha colpito tutte le classi sociali

Sarebbe un gravissimo errore considerare il voto britannico come il frutto di una decisione scriteriata.

Volete l'Europa stile Aquisgrana? L'Europa verticale? L'Europa verticistica? L'Europa fatta di assi? L'Europa intergovernativa? Quella che prevede che il Ministro tedesco faccia parte periodicamente del Consiglio dei ministri francese? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quella che dice che il Ministro francese può andare a far parte del Consiglio dei ministri tedesco? È questa l'Europa che volete? O volete l'Europa di Visegrád, un modello lontano, freddo, insensibile e incomunicabile? Quel tipo di Europa che dice: «io sto bene a casa mia, quindi non voglio nessun altro»? Questa è la seconda Europa che si prospetta.

l'euroscetticismo e il confronto tra le diversità di cultura giuridica. Infatti, qui si misura se c'è effettivamente armonia o disarmonia tra i valori, le leggi e le istituzioni. Io non ho intenzione di ritornare sul caso dei trattati internazionali, ma possiamo essere tutti d'accordo che c'è stata una prassi deviante nell'applicazione dei trattati? Penso al *fiscal compact*, che abbiamo recepito nell'articolo 81 della Costituzione che impone l'obbligo del pareggio di bilancio, ma che allo stesso tempo - ma voi tutti l'avete dimenticato - salvaguarda l'ipotesi della potestà parlamentare, che comunque resta espressione della volontà del popolo. Ma questa seconda parte del *fiscal compact* noi l'abbiamo completamente dimenticata. Per concludere, ad Aquisgrana e a Visegrád c'è solo un modello che può opporsi validamente: è il modello comunitario unitario di Roma.

Come già convenuto per le vie brevi tra i Gruppi parlamentari, le dichiarazioni di voto avranno luogo alle ore 19, con trasmissione diretta televisiva. Seguirà l'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sui più recenti sviluppi della situazione in Libia.

Signor Presidente, colleghi, nel prendere la parola non posso celare la mia commozione, oltre che il senso di frustrazione, per quanto capitato nella strada provinciale che collega la ben nota Corleone con Partinico e San Cipirello, nella quale si è consumato l'ennesimo incidente automobilistico. Questa volta

Un senso di frustrazione in quanto figura istituzionale, ma al contempo un senso di frustrazione in quanto siciliana. Credetemi, non è facile assistere alla moria dei membri della propria comunità e dei Comuni limitrofi nel percorrere la strada - ormai nota tra i miei concittadini - della morte, a seguito del lungo e perverso gioco a rimpiattino di responsabilità tra Regioni ed enti provinciali, distratti nel garantire la semplice manutenzione delle strade provinciali, che sono delle trazzere, delle trappole mortali, ovviamente anche con i riscontri negativi in termini di economia sui Comuni vicini. Il nostro Governo si è impegnato, ha inserito una norma specifica che prevede un commissario che avrà poteri sostitutivi per accelerare le procedure, in modo da poter saltare le pastoie burocratiche,

Signor Presidente, vorrei leggere alcuni passaggi di una lettera drammatica che Riccardo Morpurgo, un ingegnere di sessantaquattro anni, imprenditore edile di Senigallia, ha scritto per dire addio ai suoi cari. Si è suicidato. È un imprenditore che si è tolto la vita e che forse avrebbe potuto avere un po' più di attenzione da parte del mondo politico e del mondo giornalistico in generale, anche perché in un certo senso lo ha scritto lui stesso, laddove il senso del suo gesto drammatico potesse essere recepito come un urlo. Alcuni passaggi, però, ve li voglio leggere: «Mi sono umiliato sin dove non avrei mai creduto di dovere, potere e saper fare, ancora progettato, ancora relazionato, ancora umiliato, ho financo ipotecato il futuro mio e della mia famiglia, ed inutilmente ho ancora proposto ciò che avrebbe positivamente risolto, solo lo si fosse voluto». «Faccio scoppiare fragorosa la bomba, fiducioso che finalmente venga recepito il mio urlo, disperato». È per questo che mi permetto di leggere la sua lettera in quest'Aula. «Tanti sono gli errori che ho commesso nella mia vita (...) ma mai sono venuto meno ai dettami di correttezza ed onestà. Me ne vado dunque con la faccia pulita della persona per bene. Con il tragico, e certo insensato, gesto, spero finalmente di riuscire a risvegliare coscienze intorpidite ed animi accecati: mi rivolgo dunque ai responsabili, assolutamente irresponsabili, degli istituti di credito, ma anche ai pubblici amministratori e a chi, abusando del suo infimo potere, si arroga il diritto, tralignando la verità, di divertirsi giocando con la necessità, le ansie, le emozioni del prossimo, senza capacitarsi (FORSE) che il suo divertimento può essere recepito tragicamente da chi lo subisce, ed ancora a coloro che subiscono questa iniqua situazione avvolti nella loro assordante apatia ed indifferenza o, peggio, a coloro che la aggravano con la loro cinica e supponente cupidigia».

ha distribuito dei volantini di carattere molto volgare e triviale, con i quali invitava i ragazzi a non partecipare alla proiezione, definendo il film in maniera che qui non si può

Vorrei dirlo in maniera molto franca, Presidente, e me ne assumo la responsabilità: quel professore è indegno di rimanere professore della scuola italiana. di libertà di educazione o di libertà di pensiero, ma di capire se una persona è adeguata o meno a rivestire il ruolo di educatore e questa persona evidentemente non lo è. Due mesi fa a Basovizza, di fronte alla foiba che raccoglie migliaia e migliaia di cittadini italiani di ogni fede politica, infoibati solo perché italiani, tutte le forze politiche presenti (ed erano presenti tutte le forze politiche) hanno detto «mai più morti di serie A e di serie B», «mai più negazionismo», «mai più giustificazioni alla tragedia del confine orientale». Ma c'è qualcuno che non si arrende e non si arrende di fronte a nulla, neanche al dolore, al sangue, alle lacrime dei morti, dei loro parenti e dei loro discendenti. Non si ferma neppure di fronte alla tragedia di una povera ragazza ventenne, Norma Cossetto, che fu rapita, torturata, stuprata e infine gettata ancora viva nella foiba. Di fronte a queste persone mi domando: cosa sarebbe successo se un volantino del genere fosse stato distribuito a margine della proiezione di un film dedicato alla Shoah o alle vittime del terrorismo? Presidente, il tempo è concluso. Voglio soltanto dire che questo signore, che non voglio neanche citare perché gli darei troppa importanza, doveva scegliere se fare il professore e quindi l'educatore, oppure diventare un miserabile propagandista di odio. Credo che abbia scelto la sua strada e pertanto invito il ministro Bonisoli a cacciarlo dalla scuola italiana.

Signor Presidente, onorevoli senatori, c'è stato un disguido tra me e la Presidenza, nel pomeriggio, e non sono riuscito ad intervenire. Lo faccio adesso con parole sincere e sentite, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, per esprimere alla grande famiglia di Radio Radicale il nostro cordoglio la nostra vicinanza per la perdita di Massimo Bordin. Tanti di noi anche in quest'Aula, negli ultimi decenni hanno potuto seguire l'attività parlamentare (e non solo) attraverso la sua voce. Massimo ci ha accompagnato per anni con i suoi interventi sui quotidiani e in voce, le sue appassionati conversazioni domenicali con Marco Pannella, la sua inconfondibile rassegna stampa. Impeccabile nella panoramica quotidiana, polemica, sapientemente ironica, ma sempre caratterizzata da un punto di vista originale, espresso talvolta con un necessario commento, una chiosa sferzante, una battuta o uno di quei caratteristici e inconfondibili colpi di tosse, più o meno sofferti, che valevano quasi sempre più di un lungo editoriale. Ci mancherà questa voce, diventata ormai bandiera dell'universo radicale e pannelliano, voce e penna tagliente pure con la rubrica quotidiana che ogni giorno alimentava sulla carta stampata, non sempre condivisibile anche da parte di chi vi parla, ma tuttavia preziosa ed elemento di ricchezza per il nostro pluralismo informativo, ahimè ancora troppo carente, inadeguato rispetto alle attese dei cittadini. Ci associamo perciò alle parole della senatrice Emma Bonino con quest'ultimo ricordo e omaggio al giornalista e collega Massimo Bordin, perché ne resti in quest'Aula il prezioso ricordo e l'augurio che la terra gli sia eternamente lieve.

Senatore Rampi, non metta in difficoltà la Presidenza, altrimenti devo chiedere agli assistenti di ritirare il cartello immediatamente.

«Con molta tristezza e recriminazione devo ritirare la mia candidatura per la corsa a sindaco del Comune di Agnadello a causa di pesanti minacce ripetute nelle ultime settimane a me e alla mia famiglia». Così inizia la missiva che sta costringendo un candidato sindaco della Lega in Provincia di Cremona a rivedere la sua candidatura a pochi giorni dalla scadenza del termine elettorale. Di fronte alle sue parole non viene meno solo la candidatura di un uomo che voleva mettersi a disposizione del proprio Paese. Di fronte alle sue parole viene meno la democrazia del nostro Paese. *(Applausi Lascia spazio all'odio, alla paura, all'ignoranza di chi non prenderà mai le distanze da fatti di questo tipo, di chi si diverte a definire la Lega dispensatore di odio. di odio. Colleghi, è ora di finirla con queste inutili storie. Ditemi una volta, una sola, che qualcuno ha ricevuto danni per conto e nome della Lega! Non c'è mai stato nessun fatto del genere in tutti questi anni di politica. Non è mai accaduto! Semmai, sono state attaccate le nostre sedi: la mia, a Cremona, è stata addirittura colpita con delle bombe carta nelle settimane precedenti; ci hanno dipinto i muri; ci hanno dipinto i muri; ci hanno aggredito i gazebo. E poi noi siamo dispensatori d'odio? Noi siamo quelli che non riescono a poter mettere un candidato sindaco in un piccolo Comune di 3.800 abitanti. È questa la democrazia del 2019 del Paese Italia? Io mi vergogno di queste cose. Per andare avanti sempre su fatti del genere, quello che è successo non accade solo a uno di noi della Lega, ma a chiunque si può candidare oggi alla carica di sindaco o di assessore al proprio Comune. Io mi auguro che la questura le Forze dell'ordine intervengano e trovino subito il responsabile e che ci sia una condanna forte, pesante, a chi si macchia di gesti del genere. Poi trovarci qui e fare leggi quando i fatti sono accaduti e quando magari sono successe cose gravi, a me dispiacerebbe molto e penso anche a tutti voi. Quindi spero che la polizia faccia il suo corso, che si chiuda velocemente la vicenda e che questa persona venga messa dove deve stare: in galera.